L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***

Presidente, colleghi, come ha potuto notare chi ha assistito ai lavori dell'Assemblea, la discussione è stata molto positiva intorno ai vari pilastri di questa riforma del codice antimafia. Ricordo ai colleghi che uno dei pilastri intorno a cui si è lavorato molto, poiché abbiamo incontrato diversi problemi nel gestire a fini sociali e produttivi le aziende sequestrate e confiscate alle mafie,

licenziamenti di lavoratori e negazione dei diritti ma, all'opposto, quando interviene con misure così forti e radicali come sequestro e confisca di un'azienda lo fa perché vuole trasformare la legalità in una risorsa per creare lavoro e per migliorare la qualità dei diritti sociali presenti in quel contesto aziendale che invece la mafia negava e calpestava.

non avrà, quindi, sulle spalle un compito impossibile da raggiungere e da portare a buon fine. L'Agenzia avrà la possibilità di essere composta da 200

che devono diventare un volano di sviluppo e di promozione di diritti per molte realtà territoriali che ancora vivono un rapporto di sfiducia nel legame con le istituzioni e con il valore della legalità.

capite bene che, quando manca trasparenza proprio nella gestione dei beni confiscati, la credibilità crolla paurosamente e, quindi, anche su questo punto è stato necessario fare un salto di qualità

che gli amministratori giudiziari possano essere scelti solo per il merito, per le loro qualità professionali, per la loro autonomia e indipendenza, per essere persone in grado di poter realmente mettersi al servizio di quel bene e non di se stessi o delle cordate intorno a cui spesso si è organizzata la gestione dei beni confiscati. Colleghi, abbiamo anche previsto una serie di norme innovative, che troveranno spazio a breve nel lavoro emendativo.

per evitare quei trucchetti che abbiamo riscontrato, in base ai quali alcuni erano in grado di aggirare la soglia e quindi di poter costituire consorzi che fossero di fatto condizionati dalle imprese mafiose. stesso modo, abbiamo utilizzato l'esperienza maturata su un versante nuovo che si è spalancato di fronte a noi, che dura da anni e che ha consentito arricchimenti paurosi, addirittura ancora più consistenti di quelli che si realizzano con il traffico di deroga. Mi riferisco alle cosiddette mafie dei terreni - si pensi all'esperienza

Anche questa esperienza è servita e nel codice antimafia sono state previste norme innovative che ci consentono, anche su questo fronte, di colpire quella mafia moderna

una norma che consenta di andare sotto soglia per la certificazione antimafia, la possibilità per i parchi regionali e nazionali di utilizzare beni confiscati per farli diventare nel loro contesto una grande risorsa ecosostenibile di promozione di turismo e di agricoltura

ci consentono di sfidare questa mafia ricca, potente, violenta e pericolosa e nello stesso tempo di far diventare le risorse recuperate un'opportunità di crescita e di miglioramento della qualità dello sviluppo dei territori. Abbiamo anche potenziato una serie di norme per quanto riguarda il processo di prevenzione sia sul versante dell'efficacia, della sua modernità, sia sul versante delle garanzie. Anche questo lavoro, denso di miglioramenti, ci consente alla fine di ottenere risultati estremamente positivi. Quindi, anche questo secondo pilastro del cambiamento, dell'innovazione, è positivo e può essere ampiamente condiviso poiché consente agli operatori della giustizia di utilizzare questo strumento così delicato, e nello stesso tempo efficacissimo, tanto caro a Pio La Torre, nell'aggressione ai patrimoni, per procedere lungo questa strada e dimostrare che la ricchezza delle mafie non è più un loro punto di forza ma paradossalmente può diventare un punto di debolezza. Attraverso la ricchezza le mafie sono infatti in condizione di ottenere consenso, di riprodursi, di riorganizzarsi; ma ricevono anche colpi mortali sul piano delle sentenze penali, della reclusione più tradizionale in carcere, di quel 41*-bis* che viene confermato e che rimane uno strumento importante di tutela della dignità dei cittadini e della nostra democrazia. perché dal carcere le mafie non smettono mai, a differenza di tutti gli altri criminali, di comunicare con l'esterno, di stabilire il loro ruolo direttivo per controllare gli appalti, decidere per chi votare, condizionare l'attività economica,

delle procure e dei tribunali per quanto riguarda le misure di prevenzione. Ricordo a tutti che anche su questo punto è possibile trovare una convergenza. Poi, quando esamineremo gli emendamenti presentati potremo dare risposte adeguate, insieme al senatore Pagliari, per sbloccare alcuni intoppi che sono stati segnalati. Rimane il problema dei problemi. Ho voluto citarlo per ultimo, perché non vorrei che la discussione che ha acceso l'Assemblea e ha caratterizzato diversi interventi potesse diventare l'unica questione intorno alla quale qualificare il lavoro parlamentare. all'inserimento, fatto alla Camera, dei reati contro la pubblica amministrazione nel novero dei reati inseriti nel catalogo, insieme a quelli di mafia, di terrorismo e di altri reati associativi,

Altri, invece, hanno confermato che questa è una scelta positiva che deve essere portata avanti perché la corruzione è diventata un problema prioritario per il Paese

per estirpare, limitare ma anche superare questo fenomeno, che sta causando molti danni, soprattutto sul piano economico e patrimoniale rispetto al corretto utilizzo di risorse pubbliche,

facendo diventare sempre più severe le relative pene e facendo in modo che le Forze dell'ordine e la magistratura avessero gli strumenti più adatti per potere incidere fortemente. Naturalmente, il piano culturale, anche su questo versante, rimane un'altra leva molto importante, che, ovviamente, non deve essere messo in contrapposizione con il sistema delle norme che prevediamo sul piano penale e delle misure di prevenzione. La discussione su questo versante è aperta. C'è chi sostiene che un correttivo potrebbe aversi, ad esempio, togliendo dal novero dei reati previsti quelli che non hanno di per sé il carattere di pericolosità sociale, che - lo ricordo a tutti - è un requisito per le misure di prevenzione che rimane anche nella soluzione proposta dalla Camera e confermata in Commissione giustizia al Senato.

un altro tipo di cambiamento intorno a questi tipi di reato, cioè di legarli al carattere associativo, perché tutti i reati che fanno scattare quelle misure di prevenzione personale e patrimoniale indicate nel codice hanno questa caratteristica. Il reato di mafia è di per sé associativo, i reati di terrorismo hanno questa caratteristica; ci sono magari altri reati che non conosciamo ma che sono inseriti nel codice, come ad esempio alle associazioni sportive che esercitano violenza negli stadi, oppure, ad esempio, è prevista misura di prevenzione personale e patrimoniale per la ricostituzione del partito fascista. Insomma tutti sono collegati da questo filo che è la caratteristica associativa.

416 e non dal 416-*bis* del codice penale, in modo che il carattere di pericolosità possa reggere alla valutazione della Corte e degli organismi internazionali che hanno sempre guardato alle misure di prevenzione con molta difficoltà. Anzi, noi dobbiamo chiedere all'Europa, agli altri Paesi, di crescere su questo versante, ma lo possiamo fare se siamo in condizione di stabilire

volontà della maggioranza di mantenere sui reati di corruzione la scelta più rigorosa e ferma. Contro la corruzione, infatti, il Parlamento non può essere reticente, non può ancora una volta dare segnali sbagliati

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il lavoro compiuto

Noi eravamo di fronte al compito di fare un tagliando al codice antimafia e credo che ne sia stato fatto uno particolarmente significativo

una impostazione che possa consentire, direi oltre ai limiti del possibile, di salvare le imprese imprese sequestrate o confiscate per ragioni di mafia. In questo ambito c'è stato anche un intervento, che ritengo significativo e importante, a tutela dei lavoratori,

voglio anche ricordare rispetto al dibattito quale importanza abbia, a mio modo di vedere, aver definito il passaggio della gestione dei beni confiscati

le misure che hanno riguardato gli amministratori giudiziari, la razionalizzazione del sistema, il limite dei mandati posti agli amministratori giudiziari, che ritengo sia un limite un limite importante rispetto ad un sistema che deve garantire legalità ed etica nella stessa gestione dei

norma che potrà vedere obiettivamente il suo vero sviluppo solo quando il potenziamento del personale dell'Agenzia potrà essere realizzato

Il ruolo dell'Agenzia, che diventa centrale e portante di questo sistema, è davvero la chiave di volta rispetto alla possibilità di

il patrimonio - anche quello aziendale - frutto di attività illecite. Se questo meccanismo raggiungerà il massimo dell'efficienza e dell'efficacia, assicurando in particolare il mantenimento dei livelli occupazionali e il loro miglioramento, si realizzerà sul piano concreto la miglior forma di risarcimento dei territori

precisato. C'è una questione di fondo che credo meriti ulteriore riflessione:

e dal processo stesso di prevenzione, che è una misura straordinaria ed eccezionale che non può essere estesa indebitamente alla luce dei principi costituzionali.

voglio solo aggiungere alcune considerazioni alle repliche svolte dai relatori. Il Governo è stato impegnato fin dal primo momento nel seguire questo provvedimento

si è provveduto a individuare l'obiettivo, che è innanzitutto la gestione di un patrimonio molto ingente, rispetto al quale le risorse attualmente disponibili per l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati non sono risultate sufficienti; una maggiore razionalizzazione, l'individuazione di professionalità adeguate e la definizione di un percorso che consentisse rapidamente di mettere a valore

e, per restituirli pienamente alla società, è necessaria una corretta gestione che valorizzi tanto i beni immobili quanto, soprattutto, le aziende. Per quest'ultime la nostra maggiore preoccupazione è sempre stata quella di definire il primato dello Stato anche dal punto di vista della gestione, in modo tale che non avvenisse, dopo il sequestro o la confisca, la circostanza per la quale magari un'azienda falliva e i lavoratori, spesso incolpevoli, potessero perdere il lavoro, oltre al fatto che anche il tessuto sociale ed economico rischierebbe di essere indebolito e depauperato Sul piano normativo sono state introdotte innovazioni che sono state oggetto di considerazioni che porteranno probabilmente all'approvazione di alcuni emendamenti. Si tratta in questo senso di avere, ovviamente nel pieno rispetto del Parlamento, una volontà comune in modo tale che la convergenza di intenti, che si è determinata anche nella prima approvazione del codice antimafia, possa essere con altrettanta convergenza e capacità di intendere quale sia l'obiettivo comune. In questo senso, anche la discussione che si è

alle quali veniva sottratto un bene e sequestrata un'azienda o più attività, proprio perché il vincolo associativo doveva essere colpito, oltre alla responsabilità penale che, ovviamente, è sempre personale.

e la riqualificazione dei beni ottenuti con profitti e proventi illeciti che debbono essere pienamente restituiti alla collettività.

Presidente, preliminarmente vorrei dare atto ai signori relatori

Mi permetto, però, di non essere d'accordo con quanto proposto dal relatore - il quale sostanzialmente propone di accantonare l'articolo 1 e di passare alla votazione dell'articolo 2

proposta - vi sarà necessità di riflettere e ragionare in ordine al testo e alla possibilità di presentare o meno subemendamenti.

correttamente egli, nell'immaginare la possibilità di ancorare i reati della pubblica amministrazione a un reato associativo, ha fatto cenno all'attualità della pericolosità; ma attualità della pericolosità che - secondo il suo *in re ipsa* coperta in caso di un reato associativo e, in quanto tale, esporrebbe di meno questo provvedimento

mio avviso, signor Presidente, richiede un tempo congruo per verificare se e in che modo la modifica che i senatori relatori propongono possa o no incidere in qualche altra parte del testo. Pertanto

Signor Presidente, sulla richiesta di passare all'esame dei successivi articoli, esprimerei un parere contrario, perché l'articolo 1 costituisce innanzitutto la base del provvedimento in esame. Ed è fondamentale discutere e risolvere i problemi che esistono attorno all'articolo 1 e alla nuova formulazione che viene proposta dai relatori con la presentazione dell'emendamento 1.500. Inoltre, da un punto di vista pratico, segnalo che all'articolo 2 si fa riferimento all'articolo 1-*bis* all'articolo 5 si fa ancora riferimento allo stesso articolo. Quindi, le modifiche che potranno essere apportate all'articolo 1-*bis* costringerebbero quest'Assemblea a rinviare ulteriormente l'esame anche dell'articolo 2, dell'articolo 5 e degli altri articoli accennati. Pertanto, sarebbe più opportuno,

La seduta è tolta